la sovranità alimentare e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con riferimento all'interrogazione volta a conoscere l'attuale fase di esecuzione dei lavori di ammodernamento e rifacimento del canale Cavour, le spese già sostenute e quelle ancora da affrontare per completare l'opera, rappresento quanto segue. L'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio dell'11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito presso il Ministero delle finanze un fondo per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese, stanziando risorse per gli anni 2017-2032. del 21 luglio 2017 una parte di queste risorse sono state assegnate a questo Ministero per il periodo 2017-2021 per complessivi euro 107.654.414, di cui 92.345.169 per il rinnovo e la manutenzione della rete idrica di canali e di acquedotti e 15.309.245 per la difesa del suolo mediante interventi idrogeologici. A seguito del rifinanziamento del predetto fondo con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, il DPCM del 28 novembre 2018 ha assegnato a questo Ministero per il periodo 2018-2023 ulteriori 107.875.361 euro, destinati al settore di spesa infrastrutture anche relative alla rete idrica e alle opere di collegamento, fognature e depurazione per complessivi 215.529.775 euro. Relativamente alla ristrutturazione del canale Cavour, è stato assegnato un importo pari a 34 milioni di euro facente capo all'intervento di ristrutturazione della Rilevata Dora. Il progetto, elaborato dalle due associazioni facenti parte della Coutenza del canale Ovest Sesia di Vercelli ed Est Sesia di Novara con l'obiettivo originario di consolidare due tratte della dette Dora e Monformoso, ha registrato ritardi dovuti non solo ai tempi occorsi alle predette associazioni per acquisire l'approvazione tecnica da parte del provveditorato interregionale alle opere pubbliche, intervenuta solo nell'ottobre del 2021, ma anche per il completamento della verifica preventiva della progettazione. Sono ritardi intollerabili, pertanto sono state avviate le opportune verifiche per accertarne le responsabilità, tenendo conto che il conseguente disallineamento tra la ripartizione dei fondi stanziati in bilancio 2017-2023 e l'effettivo bisogno stimato per l'anno dall'ente ha determinato la mancata copertura di parte dell'intervento. Per tali ragioni è stato richiesto all'ente di proporre uno stralcio funzionale dell'intervento trasmesso solo lo scorso 1° marzo. I lavori previsti e finanziati con la predetta legge di bilancio del 2016 avranno quindi ad oggetto prevalentemente un intervento di restauro e ripristino della funzionalità della Rilevata Dora che interessa il fondo del canale, la struttura in muratura e i retrostanti rilevati in terra, attraverso lavorazioni da eseguirsi sia all'esterno sia all'interno del canale, al fine di assicurare condizioni di stabilità. Informo, infine, che il 30 marzo scorso, con apposito decreto, è stato concesso e finanziato sul capitolo 7470 PG1 e PG3 l'importo di 30.611.948 euro per le annualità

sé. I fondi di cui stiamo parlando sono degli anni 2016-2017, come ha spiegato lei, signor Sottosegretario, proprio gli anni del Governo Gentiloni, nei quali l'unità di missione funzionava a pieno regime. Ricordiamo che questa unità di missione è stata smantellata dal Governo gialloverde Conte I, che, come prima cosa, ha eliminato quest'unità di missione che era a Palazzo Chigi, come tale funzionava da cabina di regia e consentiva di avere una visione strategica rispetto a questi temi.

Ministeri. Tuttavia, per una mera questione di competenze all'epoca tra l'allora ministro Centinaio e l'allora ministro Costa, si decise nottetempo di farla sparire. Questo Senato ha approvato un ordine del giorno che chiede al Governo di ricreare l'unità di missione Italia sicura, che - lo ricordo veniva da un'idea di Renzo Piano. Stiamo aspettando, signor Sottosegretario, che finalmente l'unità di missione sia ricreata. Se non lo dice quest'Assemblea, lo dicono i fatti che si verificano nel Paese, con le vittime e i danni che stiamo registrando anche in questi giorni e in queste settimane. Il mio invito è quindi, in senso generale, di mettere mano a questo problema e di ricreare quella struttura che aveva fatto bene.

È un canale fondamentale, perché percorre 80 chilometri del Piemonte, dalla provincia di Torino alla provincia di Novara; è un canale che serve a irrigare le terre di un distretto risiero tra i più importanti d'Europa, vitale per la nostra economia; peraltro, chi vive in quelle terre o è coinvolto in quel settore produttivo sa bene che il canale Cavour è stato spesso spesso un'ancora di salvezza in periodi siccitosi, anche rispetto ad altre zone d'Italia dove si coltiva il riso e dove il canale Cavour non c'è. ci sono stati eventi alluvionali che hanno portato dei danni, quindi ci si aspettava che a tutti i livelli si provvedesse a sistemare quest'opera fondamentale per

però sono contento di aver portato questo tema all'attenzione del Governo. Sottolineo l'importanza che questi lavori siano completati; invito lei personalmente e quindi, tramite lei, il suo Dicastero ad assicurarsi che queste opere vengano messe in atto quanto prima, perché nell'ambito più ampio degli interventi contro il dissesto idrogeologico e le asperità ambientali, in questo caso parliamo anche di un settore produttivo fondamentale per il nostro Paese.

Italy*. Signor Presidente, onorevoli senatori interroganti, con l'atto in parola si richiedono misure specifiche per le imprese e per le cooperative a fronte degli aumenti dei costi che le stesse devono sostenere, al fine di evitare l'interruzione delle loro attività; inoltre, viene chiesto se ci sia intenzione di attivarsi in sede europea per sostenere le imprese alla luce dell'aumento dei costi di materie prime, servizi ed energia. Al riguardo, si osserva *in primis* che questo Governo è intervenuto celermente per contrastare l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, posto che, come osservato dal senatore interrogante, i citati aumenti hanno avuto pesanti ricadute sul sistema produttivo. Si ricorda, a titolo esemplificativo, che con la legge di bilancio del 2023 sono state aumentate le aliquote di credito d'imposta legato ai consumi energetici. Poiché la sfida energetica potrà essere vinta solo con investimenti e una prospettiva a lungo termine, la legge di bilancio 2023 ha previsto anche incentivi alle imprese verso investimenti in fonti di energia rinnovabile, tra i quali anche il finanziamento del fondo *green new deal* con 565 milioni di euro per il 2023, per il sostegno agli investimenti alle imprese in progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e per la transizione ecologica e l'economia circolare. Con il decreto-legge cosiddetto carburanti sono stati rafforzati i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi ed è stata istituita la commissione di allerta rapida

Il 18 maggio scorso è stato approvato alla Camera il disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto-legge bollette, che ora deve essere approvato dal Senato. Il provvedimento prevede il rafforzamento del *bonus* sociale elettrico e gas; la riduzione dell'IVA e degli oneri generali di settore del gas per il secondo trimestre del 2023; un contributo in quota fissa in caso di prezzi di gas elevati; un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas naturale; agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico. Inoltre, si ricorda che presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) è stato istituito il Fondo per il sostegno alla transizione industriale e che sono operativi i contratti di sviluppo, finalizzati a incentivare le imprese negli investimenti per la realizzazione di impianti di cogenerazione e ad alto rendimento. Le misure esposte sono rivolte all'intero sistema produttivo nel suo complesso, ivi compreso il sistema delle cooperative. Il Mimit, inoltre, ha in corso un accordo di collaborazione con Unioncamere al fine di promuovere, attraverso una rete territoriale del sistema camerale, misure di sostegno alle imprese, nonché di fornire supporto all'identificazione dell'incentivo adatto alla tipologia di cooperazione e all'investimento che l'azienda intende realizzare.

Parallelamente al monitoraggio dei costi energetici, è stato attivato presso il Mimit il tavolo tecnico sui rincari dei prezzi dei carburanti, alla presenza delle principali associazioni che compongono il CNCU e del Garante per L'obiettivo è quello di convocare in modo regolare il CNCU e le associazioni che rappresentano gli operatori del settore per affrontare i temi legati al caro prezzi, alle comunità energetiche e alle energie alternative ed operare un confronto generale sul riordino del settore. Il tavolo in parola sarà riconvocato a breve. In tale sede potranno essere senz'altro discusse le proposte avanzate da tutti gli operatori del settore, incluse quelle citate dal senatore interrogante.

si rappresenta la disponibilità ad attivarsi anche in sede europea per sostenere le imprese alla luce dell'aumento dei costi che sono chiamate a fronteggiare. ringrazio il sottosegretario Bitonci per la sua risposta. Sarò franco: trovo che non sia soddisfacente la reazione del Governo al problema enorme del caro energia che il sistema delle nostre imprese ha dovuto affrontare

Fatta salva l'estrema cortesia e gentilezza del Sottosegretario, non posso non sottolineare che la risposta a questa mia interrogazione del mese di novembre novembre arriva all'inizio del mese di giugno, quindi con molto ritardo; del resto, però, l'agire tardivo sembra essere la cifra del Governo nella risposta ai problemi sollevati dal rincaro dei prezzi dell'energia e delle materie prime, che ha messo a dura prova le nostre aziende. Le cooperative, all'interno del sistema delle imprese, hanno problemi specifici legati alle loro peculiarità. Soprattutto le cooperative sociali sono particolarmente fragili e particolarmente preziosi sono i servizi che che rendono, soprattutto alle amministrazioni locali, che appaltano attività importanti. Non c'è soltanto il problema del caro energia, rispetto al quale si è fatto troppo poco e troppo tardi. Ci sono anche altri problemi, che nell'interrogazione vengono sollevati e che vorrei nuovamente riproporre all'attenzione del sottosegretario Bitonci: quelli relativi alle basi d'asta delle gare d'appalto; quelli relativi alla necessità di immaginare forme di revisione dei prezzi finanziando l'intervento per gli appalti in corso, perché per molte cooperative lavorare con i prezzi concordati prima del caro energia sta diventando davvero impossibile. poi un'azione forte da condurre a livello europeo, che mi auguro sia sempre più vigorosa, per prevedere forme di intervento continentale a vantaggio del sistema delle aziende.

non subisca colpi che compromettano la sua possibilità di continuare a contribuire al benessere del nostro Paese e alla creazione di adeguata occupazione in Italia. Pertanto, sono insoddisfatto e in questo senso rivolgo al Sottosegretario e, per suo tramite, a tutto il Governo l'invito ad essere molto più tempestivi e molto più efficaci nel sostegno alle nostre imprese e in particolare a quelle imprese cooperative.

che fa parte dell'omonimo gruppo assicurativo controllato da Cinven partnership, tramite il fondo di *private equity* Fifth Cinven fund. Negli ultimi anni, da un'indagine condotta dall'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), sono emerse diverse problematiche di solvibilità individuale e di gruppo, nelle determinazioni delle riserve tecniche, nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, nonché in materia di gestione dei rischi e dei controlli interni. A tale circostanza ha fatto seguito un'apposita richiesta di rafforzamento patrimoniale da parte di Ivass. Tuttavia, l'azionista di controllo Cinven non ha provveduto. A partire dal terzo trimestre 2022, la capacità delle imprese del gruppo di far fronte agli impegni economici assunti si è ulteriormente deteriorata, fino a condurre alla violazione del requisito patrimoniale di solvibilità di Eurovita holding SpA e Eurovita SpA. Conseguentemente, il 31 gennaio scorso, Ivass ha nominato un commissario per la gestione provvisoria, ravvisando ragioni di assoluta urgenza, e ha sospeso le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo di Eurovita holding e Eurovita SpA, con una durata massima della gestione provvisoria fissata al 31 marzo 2023. Il 6 febbraio scorso è stato poi adottato un provvedimento di sospensione temporanea delle facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti sui contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita SpA. Eurovita SpA. Lo scopo è estremamente chiaro ed è quello di non compromettere in maniera irreversibile la situazione patrimoniale dell'impresa e ogni sua possibilità di risanamento, con con conseguente e logico grave pregiudizio per gli interessi degli aventi diritto alle prestazioni di carattere assicurativo. Come già ho avuto modo di riferire in Aula alla Camera dei deputati qualche giorno fa, il Ministro per le imprese e il *made in Italy*, su proposta dell'Ivass, ha predisposto, con decreto del 29 marzo scorso, l'amministrazione straordinaria e lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo nei confronti di Eurovita holding ed Eurovita SpA, ai sensi degli articoli 231 e 275 del codice civile. A seguito del provvedimento, l'Ivass ha nominato il commissario per la gestione straordinaria di entrambe le società e i componenti dei comitati di sorveglianza. assicurare un ordinato svolgimento dell'attività e di consentire una soluzione di mercato da parte degli organi di amministrazione straordinaria, l'Ivass ha prorogato sino al 31 giugno la sospensione dei riscatti e dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita SpA, disposta con provvedimento del 6 febbraio 2023. Rispetto alla situazione di Eurovita, l'operato dell'Ivass e delle amministrazioni coinvolte è costantemente volto alla ricerca di soluzioni finalizzate a conseguire, nel minor tempo possibile e con minor disagio possibile, la piena salvaguardia dei diritti degli assicurati e la stabilità del mercato assicurativo.

dell'Ivass, avendo anche la delega specifica, ho informato subito il Ministro, che ha provveduto in maniera estremamente celere

mercato. Dalle notizie e dalle informazioni che abbiamo, si sta andando verso una soluzione che ovviamente deve tener conto della tutela degli assicurati, ma anche - ciò è estremamente chiaro ed evidente - della tutela dei consumatori e dei risparmi di chi

effettuati dalle compagnie assicurative. La variazione dei tassi e quindi dei rendimenti ha minato in maniera molto evidente, in questo come anche in altri casi di carattere internazionale (se guardiamo al di là dell'oceano), la possibilità da parte

non abbiamo ancora una risposta, nel senso che ci sono circa 400.000 clienti di Eurovita in attesa. Si calcola che i riscatti potrebbero riguardare 350.000 di loro (parliamo di 10 miliardi di di euro di risparmi). Ricordiamo tutti che, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, la tutela del risparmio è un valore, perché l'Italia è una

Quello che capiamo di questa vicenda è che tale assicurazione (Eurovita) e il suo azionista di maggioranza non sono stati in grado di rassicurare l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni sulla propria

al momento non vediamo. Capisco bene le sue osservazioni: fa riferimento all'aumento dei tassi e quindi alla difficoltà, non solo per gli istituti gli istituti assicurativi, ma anche per quelli bancari, di far fronte a questa nuova situazione internazionale, che è molto cambiata rispetto ai decenni nei quali ci siamo abituati a tassi vicini allo zero, se non addirittura negativi. Infatti, come lei giustamente ha detto, le crisi bancarie che abbiamo visto accadere, in particolare dall'altra parte dell'oceano (ma sappiamo che anche in Europa ci sono stati problemi),

che consentano alle imprese di tornare sul mercato. Mi sembra di capire che si parla di 250-300 milioni di capitale: questa è la somma che bisognerebbe trovare, che non è banale, naturalmente. Bisogna trovare una soluzione:

lasci fare una digressione, che ha a che fare con un'altra questione che abbiamo sul tavolo, strettamente collegata. Se lei e io infatti stiamo qui a discutere di tutela del risparmio, di crisi di fiducia dei mercati e di difficoltà di chi gestisce il risparmio

che, come sappiamo, crea quel *backstop* - quindi un meccanismo di gestione di eventuali crisi bancarie - che farebbe bene soprattutto al nostro Paese. Le Le banche italiane sono solide - anche il governatore Visco ha detto che il sistema bancario è solido - ma sappiamo che il nostro listino borsistico è pieno di titoli bancari e, quando c'è una crisi di fiducia rispetto al risparmio gestito, delle banche in particolare, e si verifica una crisi in Svizzera o in California, il listino di Milano è il primo a precipitare, dal momento che viviamo in un meccanismo interconnesso e complesso, per cui dovrebbe essere considerato interesse nazionale il fatto di avere un sistema sovranazionale che blocca le crisi bancarie.

tratta di una responsabilità gravissima, signor Sottosegretario, perché, se oggi avessimo quel meccanismo funzionante, saremmo tutti più tranquilli, i nostri risparmiatori e il Paese sarebbero più tranquilli, ma per ragioni ideologiche non vediamo ancora questa ratifica. Scommetto che prima o poi arriverà e sarà una delle molte cose su cui avete cambiato idea, ma speriamo che accada prima piuttosto che dopo.

collega Malpezzi per la possibilità che mi offre di comunicare che il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è ormai giunto in dirittura d'arrivo. A seguito di una lunga interlocuzione con la Commissione europea, siamo infatti addivenuti a un nuovo testo, anch'esso pienamente condiviso con il Ministero dell'università e della ricerca e ora sottoposto alle definitive valutazioni della stessa Commissione. L'impostazione attuale del DPCM intende valorizzare, ai fini dell'uniformità dei percorsi, sia i contenuti professionali minimi del docente, sia il ruolo di garanzia svolto dall'Agenzia nazionale di che costituisce il principale presidio dell'omogeneità dei requisiti qualitativi dell'offerta formativa. In merito ai contenuti specifici del DPCM, preciso che al momento non si rende possibile entrare nel dettaglio, in quanto il testo, come già detto in precedenza, dev'essere prima validato, quanto meno nella sua nuova impostazione generale, dalla Commissione europea. In ogni caso, posso anticipare fin d'ora che il DPCM individua puntualmente: i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e solidità; le modalità di organizzazione degli stessi al fine di realizzare una collaborazione strutturata e paritetica tra sistema scolastico e istituzioni della formazione superiore; i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa dei percorsi, con l'obiettivo di assicurare un'erogazione uniforme ed omogenea su tutto il territorio nazionale, nonché gli eventuali costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale che tengono conto delle diverse tipologie di partecipanti. Infine, mi preme segnalare che l'adozione del DPCM non esaurirà le azioni di questo Governo per favorire l'attuazione della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista dal PNRR e definita nella precedente legislatura. Infatti, proprio al fine di meglio regolare talune delle questioni citate dal presente atto ispettivo - mi riferisco in particolare alle modalità di erogazione della didattica e alla definizione di strumenti di flessibilità organizzativa al fine ultimo di accrescere al massimo la disponibilità dell'offerta formativa da parte dell'università - preciso che vi è la necessità di intervenire su talune previsioni normative della riforma rivelatesi non coerenti con il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Si tratta di correttivi che stiamo proponendo in sede di conversione del decreto-legge cosiddetto e che, se approvati, potranno contribuire positivamente, sia ad ampliare l'offerta formativa dell'università, sia a ridurre i costi di erogazione dei percorsi, a beneficio finale degli aspiranti docenti della scuola.

quasi simile a quella che il Ministero ha dato nell'altro ramo del Parlamento circa due settimane fa. Dico quasi simile, ma non risolve le questioni che abbiamo sollevato e che ci stanno particolarmente a cuore per una serie di elementi. Provo a metterli in ordine, consegnandoglieli, Sottosegretaria, in modo tale che possa a sua volta consegnarli al Ministro per poter dare una risposta, se non al Partito Democratico, agli studenti e alle università. Quali sono questi elementi? Primo: le università e gli studenti, che non sono stati ancora coinvolti con le loro rappresentanze studentesche, non hanno alcun tipo di indicazione circa il percorso dei 60 CFU (crediti formativi universitari), perché non ne conoscono i contenuti. Quindi, non hanno idea né le università, né i rappresentanti degli studenti di quale direzione intraprendere, anche a livello organizzativo. siamo in grandissimo ritardo, perché sappiamo anche noi che c'è una data di scadenza ben precisa, che le 70.000 assunzioni dei nuovi insegnanti devono avvenire entro il 2024 e che si deve correre. Per ora il percorso è ancora tutto tutto molto indefinito e - come ricordava giustamente lei - è un percorso che è stato legiferato nel decreto-legge n. 36 del 2022, esattamente un anno fa, ma non sono più partiti i decreti attuativi. Stiamo ancora aspettando e non abbiamo chiarimenti.

costi. Noi come Partito Democratico in quella sede di conversione avevamo chiesto che venisse inserito lo stesso sistema che si utilizza per l'università, e cioè ampliare la cosiddetta *no tax area*, spostarla anche in quell'ambito, in modo tale da essere sicuri che gli studenti potessero accedere a quel tipo di percorsi in modalità sostenibile. In caso contrario, si parla di costi - lo riportano le fonti di stampa, ma mi aspetto che il Ministero possa chiarire che possono arrivare a 2.500 euro. Non è possibile dire ai nostri ragazzi che vogliono diventare insegnanti che quel percorso lo devono pagare loro. Quindi,

che metteva un massimo di costi per quelli che erano allora i 24 crediti, che era fissato in 500 euro - una sorta di contributo, ma per il resto ci pensa lo Stato - altrimenti così non può funzionare. Noi vediamo anche il messaggio della *no tax area*, che quindi riguarda l'ISEE e potrebbe avere un significato all'interno del Piano per il diritto allo studio e in questo modo essere riconosciuto. C'è un altro elemento che ci preoccupa: siccome comprendiamo che c'è un ritardo, noi sapevamo che all'interno di quel decreto c'era una quota di erogazione della formazione *online;*

di questi percorsi c'è una parte importante di tirocinio, perché i nostri futuri insegnanti non devono solo avere le competenze - le conoscenze dovrebbero essere già certificate - ma devono anche saperle trasmettere. Quindi, era necessario anche il tirocinio. È È vera la notizia che questa percentuale di formazione erogata *online* può essere aumentata, addirittura al 50

chiarezza e una compartecipazione. Non volete confrontarvi? Il Ministero non vuole confrontarsi con le Commissioni competenti perché non è tenuto in maniera così netta? Bene: lo faccia con le università e con le rappresentanze studentesche. Abbiamo bisogno

alle quali risponderanno il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'istruzione e del merito. Il senatore Magni

finestra") sulle procedure di valutazione di economicità, efficienza ed efficacia nell'impiego dei fondi del PNRR, Signor Presidente, signor Ministro, la stampa ha reso noto nel mese di maggio che la Corte dei Conti ha evidenziato ben due volte criticità relative all'attuazione dei progetti del PNRR. il 3 maggio, in sede di controllo concomitante, ha messo in luce rilevanti criticità sui traguardi previsti per il semestre in corso. In particolare, la Corte ha sostenuto il mancato conseguimento del *milestone* comunitario che chiedeva di aggiudicare, entro il 31 marzo scorso, gli appalti per almeno quaranta stazioni di rifornimento ad idrogeno per il trasporto stradale e ha definito, in sostanza, che siamo di fronte a un grave ritardo, ormai consolidato, prodotto da un generale difetto di programmazione. L'obiettivo è di aggiudicare, quindi, entro il 30 giugno, i lavori per le colonnine per per le colonnine per ricaricare i veicoli elettrici nelle autostrade e nelle aree urbane. In secondo luogo, la Corte ha posto che tali criticità possono essere quantificabili quali gravi irregolarità gestionali ai fini della responsabilità dirigenziale. In seguito, il 25 maggio, la Corte ha pubblicato un rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, nel quale si evidenzia come il Piano abbia finora portato un impegno di risorse decisamente inferiore rispetto a quello annunciato. I conti evidenziano come, nei primi quattro mesi del 2023, erano stati spesi 1,1 miliardi, su una programmazione di 32,7 miliardi per l'intero 2023. Abbiamo letto alcune dichiarazioni molto contrariate, sue e del suo Sottosegretario.

controllo sui fondi del PNRR e, dall'altra, di intervenire limitando la punibilità di amministratori e dipendenti pubblici, ignorando pesanti critiche avanzate sul punto dal Presidente della Corte dei Conti durante il discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

dai Ministeri, che non hanno i fondi per stabilizzarli e voi non avete previsto di finanziarli. Questo non può che confermare, in modo grave, la situazione di difficoltà organizzativa e gestionale

per stabilizzare realmente gli esperti impegnati nel PNRR e di promuovere una leale collaborazione tra gli organi costituzionali in vista dell'obiettivo

le riforme e gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel corso di questi mesi, il Governo ha provveduto a effettuare una verifica approfondita di cui si darà conto nella terza relazione approvata proprio ieri dalla cabina di regia e della quale ha preso atto il Consiglio dei ministri, che verrà inviata nei prossimi giorni per un dettagliato dibattito che sicuramente avverrà all'interno del Parlamento. Si tratta di una verifica effettuata nella prospettiva di garantire, da un lato, un utilizzo efficace di tutte le risorse e dall'altro, di individuare in relazione a tutti gli investimenti le modalità di attuazione, le forme di finanziamento più adeguate rispetto agli obiettivi e la loro effettiva realizzazione. In questo contesto, si inseriscono anche le possibilità che sono state offerte dal regolamento REPowerEU, che rappresenta un'ulteriore sfida per l'Italia sia dal punto di vista della tempistica sia della numerosità degli investimenti finanziabili. Quanto alla presunta intenzione del Governo di limitare le competenze e il ruolo della Corte dei conti, evidenzio che la situazione è molto diversa da quella illustrata dagli interroganti. L'articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, ovvero la disposizione che, al fine di superare la cosiddetta paura della firma, limita la responsabilità erariale per le condotte omissive ai soli casi di dolo, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico dal secondo Governo Conte quale risposta alla necessità di favorire la ripresa economica post-Covid. La medesima disposizione è stata prorogata fino al 30 giugno 2023 dal Governo Draghi per favorire l'attuazione del PNRR e del Piano L'emendamento governativo depositato ieri alla Camera dei deputati in relazione al disegno di legge n. 44 si limita esclusivamente a prorogare quanto deciso dal Governo Conte e prorogato dal Governo Draghi. Pertanto, si tratta di un'iniziativa assunta dall'attuale Esecutivo al pari dei precedenti quale risposta transitoria e parziale rispetto a una più ampia esigenza di intervento riformatore in materia di responsabilità amministrativo-contabile. Quanto all'attività di controllo della Corte dei conti in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza, evidenzio che il controllo concomitante della Corte è stato previsto dall'articolo 11 della legge n. 15 del 2009 ed è rimasto inattuato per oltre un decennio, ovvero fino alla decisione assunta con la legge n. 76 del 2020. Dunque, la previsione del controllo concomitante non nasce per il PNRR, che all'epoca neppure esisteva. Relativamente al PNRR, invece, la disciplina specifica sul controllo della Corte dei conti è da trovarsi nell'articolo 7 del decreto-legge n. 77 approvato durante il Governo Draghi. In particolare, detta disposizione affida alla Corte dei conti il controllo dei fondi del PNRR nella modalità del controllo successivo sulla gestione e non di quello del controllo concomitante. In attuazione dell'articolo 22 della legge n. 76, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha varato un'organizzazione del Collegio del controllo concomitante presso la sezione del controllo successivo della gestione delle amministrazioni centrali dello Stato. Tale delibera istituiva questo organismo senza far riferimento alla legge n. 77 del 2001. In conclusione, nonostante questo, il Governo ha messo in campo e vuole attuare una politica di coordinamento nel lavoro con la Corte dei conti anche per quanto riguarda l'attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 77 del precedente Governo. L'attività della Corte dei conti in materia di PNRR è chiaramente disciplinata dal decreto n. 77 e non c'è alcuna intenzione di intervenire su quanto in esso è previsto. Questa è una ricostruzione corretta dal punto di vista legislativo della tempistica delle questioni di cui oggi ci occupiamo.

quindi arrabbiare, si può anche non essere d'accordo e la politica può fare altre scelte, però certamente tali istituzioni hanno una loro autonomia ed è giusto che diano la loro valutazione e i loro giudizi. Lei stesso

Avete il diritto di governare, perché il popolo vi ha dato la maggioranza per farlo, ma non di mettere in discussione gli organi di controllo, che sono autonomi e rappresentano l'insieme degli italiani e del Parlamento.

iniziale dovrebbero essere presentati entro il 30 aprile, quindi siamo in ritardo. Il Ministro ci ha fatto sapere più volte che c'è la data di fine agosto, ma quella è la data ultima, quindi siamo molto preoccupati che si accumulino ritardi su ritardi e che non scattino risorse anche della programmazione precedente che possono essere utilizzate.

Noi siamo decisamente contrari e chiediamo se il Governo intenda utilizzare i fondi del PNRR o fondi di coesione, prendendo quindi risorse da progetti che sono originariamente definiti sul PNRR e spostandole su

per scelte importanti come quelle di sostegno al Governo ucraino per il diritto alla legittima difesa, penso non ce ne sia davvero bisogno, ma vogliamo sapere se il Governo intenda avvalersi di quella facoltà a cui siamo decisamente contrari. Signor Presidente, vengono poste diverse questioni contemporaneamente, quindi farò una sintesi delle tre per dire che l'Italia sta seguendo esattamente il percorso che stanno seguendo tutti gli altri Stati membri. Vorrei ricordare che ad oggi sono solo cinque i Paesi europei che hanno presentato le modifiche del loro Piano nazionale di ripresa e resilienza insieme al REPowerEU, quindi non c'è alcun ritardo da nessuna parte. Soprattutto, in una comparazione con gli altri Paesi europei si può intravedere, come emergerà in modo molto dettagliato dalla relazione che abbiamo presentato, che non esiste un ritardo, ma ci sono un dialogo e un confronto costanti con la Commissione europea rispetto agli obiettivi da realizzare all'interno di questa modifica. Tali obiettivi partono da un dato, il primo, che è collegato alla presentazione del capitolo aggiuntivo REPowerEU, per il quale il Governo ha per tempo avviato un tavolo unico con tutti i soggetti interessati, a partire dalle parti sociali e dalle organizzazioni datoriali, ma anche e soprattutto con le principali aziende di Stato interessate, per poter costruire

Abbiamo già individuato la possibilità di avere risposte preventive sull'ammissibilità o meno degli interventi, perché questo ci consente di avere preventivamente un quadro che si definirà con la presentazione del programma REPowerEU in forma aggiuntiva, come capitolo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei termini previsti da regolamento, ossia il 31 agosto di quest'anno. Questo dice il regolamento; può anche non piacere, ma è così. L'ultima considerazione è collegata alla richiesta specifica sulla questione relativa al regolamento della Commissione europea per la produzione di munizioni (ASAP), sulla quale proprio oggi il Parlamento europeo si è espresso. Abbiamo già detto - ma lo voglio ribadire in modo molto chiaro - che il sostegno non è in discussione. La facoltà di accedere all'utilizzo di quelle risorse a tale scopo, per quanto riguarda questo Governo, non è in alcun modo all'ordine del giorno. PRESIDENTE.

dei progetti modificati. Ad ogni modo, ci torneremo in Aula presto, perché abbiamo chiesto di confrontarci con la maggioranza con uno specifico atto indirizzo. Signor Ministro, oggi a Bruxelles il Gruppo dei Socialisti e Democratici ha presentato, su iniziativa del Partito Democratico e della delegazione italiana, emendamenti che prevedevano espressamente l'eliminazione della possibilità di utilizzo, attraverso i fondi del PNRR, di risorse per l'acquisto di armi e munizioni - gliela dico così perché questa è la sostanza - ma sono stati respinti e affossati dai suoi colleghi nel Parlamento europeo. Infatti, i deputati del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, di Identità e Democrazia e del Partito Popolare Europeo hanno votato contro. Quindi, signor Ministro, noi dovremmo fidarci della sua parola, ma oggi nella seduta plenaria del Parlamento europeo è andata in scena esattamente un'azione opposta a quella che lei ha riferito qui. Con il voto dei Gruppi appartenenti al centrodestra italiano, oggi sono stati affossati emendamenti che ci avrebbero garantito che quelle risorse non sarebbero mai state utilizzate a tal fine. Ricordo a tutti noi che il PNRR lo abbiamo ottenuto per ridurre le diseguaglianze, i divari territoriali, generazionali e di genere e soprattutto per rafforzare scuola, sanità, trasporti, transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale. Signor Ministro, è necessario votare su questo no. Non ci bastano le sue parole. ci bastano le sue parole. È evidente che il voto a favore di questa possibilità espresso oggi dai Gruppi di centrodestra presenti nel Parlamento europeo ci preoccupa. Ragion per cui, signor Presidente, il Partito Democratico conferma la necessità di votare al più presto un atto di indirizzo che trasformi l'impegno del ministro Fitto in atti non più reversibili.

Signor Presidente, signor Ministro, per l'attuazione del PNNR sono stati riconosciuti all'Italia 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti, erogarsi in dieci rate subordinate al raggiungimento di specifici obiettivi qualitativi e quantitativi indicati nel medesimo PNRR. Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli eventi geopolitici senza precedenti provocati dalla guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina e l'aggravarsi delle conseguenze dirette e indirette della crisi del Covid-19 hanno avuto rilevantissime ripercussioni sulla società e sull'economia dell'Unione, sulla sua popolazione e sulla coesione economica, sociale e territoriale. Il 18 maggio 2022, la Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU, che rappresenta la risposta dell'Unione europea alle perturbazioni del mercato energetico globale causate dall'invasione russa dell'Ucraina. In data 1o marzo 2023, è entrato in vigore il regolamento n. 435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che, nel modificare il regolamento n. 241 del 2021, prevede l'inserimento nel PNRR del capitolo dedicato al piano REPowerEU L'iniziativa REPowerEU è stata attuata dalla Commissione europea anche mediante l'introduzione di opportune modifiche ai programmi legate alle politiche di coesione, allo scopo di renderli idonei a fronteggiare l'emergenza energetica. Al regolamento REPowerEU, infatti, è collegata la possibilità di utilizzare le risorse della programmazione 2014-2020 per finanziare misure eccezionali, al fine di supportare le piccole e medie imprese colpite dall'aumento del prezzo dell'energia e sostenere le famiglie bisognose nell'affrontare le spese energetiche, unitamente all'uso flessibile del Fondo europeo di sviluppo regionale e dei Fondi strutturali europei. Pertanto, l'introduzione del capitolo aggiuntivo PNRR relativo a REPowerEU consente di avviare l'allineamento dei quadri programmatori delle diverse fonti di finanziamento, sia europee sia nazionali, in materia di coesione e di assicurarne il coordinamento per una gestione maggiormente efficace ed efficiente. Avendo l'Italia già utilizzato tutta la quota dei contributi a fondo perduto di 122 miliardi di euro, sotto forma di prestiti resi disponibili dal dispositivo di ripresa e resilienza, la quota italiana dei fondi di REPowerEU è pari a 2,7 miliardi di euro, ai quali si può aggiungere fino al 7,5 per cento dei fondi relativi alla programmazione 2021-2027 della politica di coesione. È indispensabile che il capitolo REPowerEU del PNRR italiano sia costituito da riforme e investimenti non solo realizzabili entro l'arco temporale del dispositivo di ripresa di resilienza, ma anche in grado di contribuire effettivamente a realizzare gli obiettivi di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili,

il Governo ha comunicato di aver avviato, così come previsto dalla comunicazione della Commissione europea, pubblicata in data 3 marzo 2023 e recante gli "Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU", costanti interlocuzioni con la Commissione europea in ordine all'avanzamento dell'istruttoria relativa all'aggiornamento del PNRR e al capitolo REPowerEU. Si chiede quindi di sapere quali sono le iniziative assunte a livello nazionale ed europeo dal Governo relativamente alla definizione del capitolo REPowerEU all'interno del PNRR italiano. PRESIDENTE. Il ministro

uno dei punti centrali dell'azione relativa alla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo dico anche collegandomi alle ragioni di carattere esterno che hanno determinato la definizione del regolamento REPower da parte della della Commissione europea, successivamente all'invasione dell'Ucraina e alle conseguenze della crisi energetica che ne sono derivate. In modo particolare vorrei ricordare, proprio per dare una risposta strutturale, che il Governo, nella sua prima legge finanziaria, su 35 miliardi di euro disponibili, ne ha dovuti mettere a disposizione 21 per andare incontro all'aumento del costo delle bollette per famiglie ed imprese. È evidente quindi che il tema del REPower assume per diversi aspetti una rilevanza particolare. Il primo è collegato al fatto che vi è la necessità di rafforzare l'autonomia strategica del nostro Paese. Il presidente del Consiglio Meloni lo ha fatto in un incontro specifico con i vertici di ENI, Enel, Snam e Terna, mettendo in campo una definizione degli interventi dal punto di vista del rafforzamento della rete. Al tempo stesso, si sta lavorando in modo coordinato con tutti i Ministeri interessati per costruire una misura di interventi sul fronte degli incentivi che sia in grado di dare una risposta all'efficientamento energetico per famiglie e imprese. Allo stesso modo, nella cabina di regia, così come modificata dal decreto-legge n. 13 del 2023 sulla *governance*, che ha attribuito un ruolo particolarmente rilevante e fondamentale alle parti sociali e alle organizzazioni datoriali, si sta lavorando per condividere i contenuti del REPowerEU, al quale - come è stato ricordato

delle risorse utilizzate dalla politica di coesione. Su questo lavoro abbiamo messo in campo un'iniziativa nel rapporto con le Regioni, che si sta sviluppando anche grazie a incontri con i singoli Presidenti di Regione, per definire un coordinamento tra le risorse del PNRR e quelle della coesione, essendo due programmazioni che il Governo ha deciso sin dall'inizio di coordinare in modo organico. All'interno di questo, nei prossimi giorni, sarà definito il quadro di riferimento sia finanziario complessivo sia dal punto di vista dei singoli interventi e non mancherà la possibilità di discuterne in Parlamento, come questo Governo ha sempre fatto su questo tema sin dall'inizio della legislatura.

soddisfatto, e per gli impegni e per la competenza che profonde nel difficile compito di dare concretezza alla rimodulazione della spesa del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare ai fini di ottimizzare le sinergie delle risorse destinate a un settore strategico come quello energetico.

il PNRR ha stanziato per asili nido e scuole per l'infanzia circa 4 miliardi di euro per interventi infrastrutturali e circa un miliardo per il potenziamento dei servizi nella fascia di età da L'obiettivo è garantire alle famiglie italiane oltre 260.000 nuovi posti negli asili nidi. Sono numeri importanti. Qualche giorno fa si sono svolti gli stati generali della natalità, alla presenza di Sua Santità Papa Francesco. I figli sono un investimento per il bene comune, senza di loro una comunità non ha futuro. Noi siamo qui oggi per dire con forza che credere nel valore della natalità vuol dire investire sulle politiche di conciliazione lavoro-famiglia e sul *welfare* familiare.

deve arrivare dai fondi del PNRR. Ecco perché oggi pomeriggio pongo tale questione all'attenzione del ministro Giuseppe Valditara, che ringrazio e che so essere molto attento e sensibile su questi argomenti. L'investimento del PNRR su asili nido e scuole dell'infanzia è un obiettivo che il nostro Paese non può mancare, come lei ha giustamente sottolineato più volte, signor Ministro. Penso ad esempio al Veneto, dove una novantina di progetti sono stati ammessi al finanziamento per quasi 200 milioni di euro

esecutiva per la realizzazione dei progetti del PNRR sono state riscontrate delle problematiche da parte degli enti territoriali, in modo particolare dai Comuni più piccoli. A questo aspetto si aggiunge anche un altro importante fattore: l'aumento dei prezzi dei materiali, che si è tradotto in un ostacolo significativo per le stazioni Ecco perché oggi in quest'Aula vorrei chiederle se non intenda prorogare i termini delle procedure di assegnazione dei lavori, per dare risposte positive ai Comuni sugli eventuali ritardi nell'esecuzione dei progetti, e se corrisponde al vero - come ho appreso da fonti di stampa l'intenzione di ridurre le risorse stanziate per la realizzazione di scuole dell'infanzia e asili nido.

Signor Presidente, gentili senatori, è ferma intenzione del Governo fare in modo che tutti i fondi messi a disposizione dall'Unione europea siano spesi nel modo più efficace, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR. Dobbiamo tuttavia prendere atto che il mutato scenario economico ci ha imposto di rivedere le strategie per rispettare le scadenze del PNRR e garantire al tempo stesso la qualità e la sostenibilità dei risultati. L'aumento dei costi dell'edilizia, stimato del 30 per cento, ha un impatto oggettivo sugli obiettivi che possiamo realizzare con le risorse del PNRR. È doveroso dunque precisare che, in vista della revisione del PNRR, contrariamente a quanto è stato affermato da qualche parte in questi giorni, non abbiamo previsto alcun taglio alle risorse, ma solamente una rimodulazione degli obiettivi, al solo fine di renderli compatibili con le risorse assegnate, che sono sempre le stesse, ed evitare di perdere i finanziamenti europei. Ricordo inoltre che, al fine di colmare i ritardi connessi alla realizzazione del Piano asili, un primo passo in questa direzione è stato fatto con l'ultimo decreto PNRR, con il quale siamo intervenuti con un pacchetto di semplificazioni amministrative davvero eccezionale, che ha consentito una forte accelerazione degli interventi in materia di edilizia scolastica semplificazioni modellate sul cosiddetto modello Genova. I primi riscontri, che ci vengono anche da interlocuzioni con l'Unione delle province d'Italia (UPI) e con ANCI, sono confortanti. In particolare, proprio al fine di rispettare le tempistiche indicate, è stata riconosciuta ai sindaci e ai Presidenti di Province e di Città metropolitane la possibilità di operare come commissari straordinari, nonché di avvalersi di specifico supporto tecnico, anche esterno alle proprie amministrazioni. Quest'ultima disposizione favorisce specificamente gli enti locali di minori dimensioni, i quali non sempre hanno nel proprio apparato le professionalità tecniche necessarie per seguire lo svolgimento degli appalti. Da ultimo rappresento che il Ministero, con l'avviso pubblico del 10 maggio scorso, ha prorogato al 20 giugno 2023 il termine per l'aggiudicazione di lavori inizialmente fissato al 31 maggio 2023, in tal modo riconoscendo ulteriore tempo per la conclusione delle procedure amministrative a beneficio dei Comuni. Quanto fin qui illustrato dimostra che, ben diversamente da chi ritiene che sia stato proposto un taglio di risorse, stiamo invece lavorando con determinazione per gestire in maniera sinergica ed efficiente tutte quelle messe a disposizione, alle quali peraltro abbiamo aggiunto proprio nel settore dell'edilizia scolastica ulteriori 1,2 miliardi di euro non PNRR e non preventivati dal precedente Governo. intervenire in replica il senatore De Poli, per due minuti. Le sue parole ci confermano che sui temi della natalità, del *welfare* familiare e delle politiche per la conciliazione tra lavoro e famiglia Governo e maggioranza stanno lavorando concretamente per invertire la rotta. sono però soprattutto i cittadini a casa, le comunità e i nostri territori. Abbiamo il dovere di utilizzare, come lei ha detto, tutte le risorse del PNRR e metterle a terra. Quindi la proroga prevista per gli interventi ulteriori è fondamentale per dare queste risposte e questo è un obiettivo che il Governo sta perseguendo con il massimo impegno, così come in modo particolare il Ministero da lei guidato. Vorrei anche ringraziare tutta tutta la struttura amministrativa, che credo in questi giorni abbia migliaia e migliaia di richieste da parte degli enti locali, in modo particolare chiaramente quella che segue tutti i lavori del PNRR, perché non è facile, visto che ognuno ha la sua peculiarità e il suo problema e in questi giorni è investita da mille

la mattina del 29 maggio uno studente di sedici anni, che frequenta un istituto di istruzione superiore di Abbiategrasso, in Provincia di Milano, ha aggredito con un coltello una delle sue professoresse in classe, durante l'orario di lezione, con conseguente *shock* anche dei suoi compagni. Com'è noto, l'insegnante ha riportato un taglio a un braccio e altre ferite più lievi ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano, dov'è ancora ricoverata. L'episodio, di evidente e oggettiva gravità, è anche espressione di un malessere purtroppo assai diffuso tra i giovani del nostro Paese. Sempre più studi e analisi concordano sul fatto che questo malessere sia stato anche anche acuito dal lungo isolamento domestico dovuto alla pandemia. Questo atto ritengo che debba spingere tutti noi e l'intera comunità nazionale a riflettere sulle ragioni più profonde che possono portare a gesti così estremi, ma reputo anche che l'introduzione della figura del docente *tutor* o dello psicologo, signor Ministro, forse non sia davvero sufficiente. Servono sicuramente più fondi per rafforzare queste figure, ma anche se vogliamo maggiori interventi sul piano culturale, a maggior ragione in un contesto *post* pandemico che - com'è evidente - ha incrementato l'utilizzo dei *social*, il cui abuso o cattivo utilizzo non incide positivamente sulle vite dei ragazzi. Sono giovani il

che purtroppo nell'ultimo decennio evidentemente è venuto meno. Quindi, con questa interrogazione, signor Ministro, le chiediamo, per quanto di sua competenza, come intenda intervenire concretamente, ma anche con urgenza, per arginare e ancor di più prevenire fenomeni di violenza sempre più numerosi, al di là del caso specifico, e che sono di una gravità quasi intollerabile, che - lo confesso -preoccupa non poco.

da cui mi ero subito recato per comprenderne personalmente le condizioni. Al di là della gravità e specificità di questo episodio, affiora - com'è stato giustamente sottolineato - un diffuso malessere nei giovani, acuito da ultimo dal contesto pandemico e dal conseguente confinamento che ha interrotto la relazione interpersonale, che è fondamentale nello sviluppo educativo. Credo profondamente nella scuola proprio come comunità umana ed educante, che appunto strategica per lo sviluppo anche psicologico dei nostri ragazzi. A fronte di questo quadro, credo che occorra innanzitutto ricreare nella scuola un clima di serenità per valorizzare proprio quella comunità educante impegnata ogni giorno a sostenere e sviluppare i talenti di ogni ragazzo, ponendo particolare attenzione alla personalità del singolo, perché viva il suo processo di crescita senza che questo generi situazioni conflittuali. Va pertanto visto con favore il rafforzamento di forme di sostegno psicologico a favore della comunità scolastica, soprattutto per gli studenti che manifestino particolari forme di disagio. A tal riguardo lavoreremo, insieme con il Ministero della salute e ovviamente con il Parlamento, presso il quale già insistono diverse proposte di legge, affinché vengano definite soluzioni di sistema e non episodiche come quelle disposte in seguito alla pandemia. Ho inoltre convocato le associazioni dei genitori, cui ho chiesto di discutere insieme a noi misure per costruire quella grande alleanza che deve unire famiglie, docenti, studenti e mondo della scuola in generale. Al fine di intervenire in modo efficace su alcune manifestazioni specifiche di questo disagio, è innanzitutto necessario avere un quadro preciso del fenomeno. Per questo motivo, ben prima di quest'ultimo episodio, avevamo già deciso di realizzare sia il tavolo di lavoro per affrontare i temi del bullismo a scuola, sia una specifica banca dati per comprendere i reali numeri dell'aggressione ai docenti e al personale della scuola. È chiaro che la delicatezza e la diffusione della problematica richiedono una molteplicità di azioni, molte delle quali sono già in essere, tutte convergenti al fine di intercettare e arginare comportamenti a rischio da parte degli studenti. Anche la personalizzazione della didattica a cui lei faceva riferimento - cosa di cui la ringrazio - che abbiamo voluto incarnare nella figura del docente *tutor* e del docente orientatore può certamente dare un contributo importante. Tra queste rientra, appunto, l'investimento che stiamo mettendo in atto per il percorso di personalizzazione, che a mio avviso è strategico. Signor Presidente, signor Ministro, quello che è accaduto è un episodio che naturalmente dev'essere circostanziato, nel caso specifico, in quella condizione specifica, familiare e umana, ma non può non essere la spia di un malessere che, come giustamente veniva ricordato, è diffuso tra i nostri ragazzi.

il fatto che lei non abbia citato altre due questioni che abbiamo trattato in questa interrogazione e alle quali teniamo moltissimo. Avete avuto una responsabilità abbastanza pesante nel nel destrutturare l'intervento 18app, che era un investimento sui nostri ragazzi. Ebbene, credo che questo sia un elemento su cui dovete riflettere necessariamente, perché

di studi negli "ITS Academy" in modo che questi istituti tecnici superiori costituiscano la formazione terziaria, ma non universitaria, che dovrebbe rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione,

le sei aree tecnologiche dei corsi di durata biennale o triennale sono: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il *made in Italy* (sistema agroalimentare, sistema casa, sistema meccanica, sistema moda, servizi alle imprese), tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turismo, tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Sappiamo che lei, signor Ministro, sta lavorando molto su questo ulteriore percorso di studi, per il quale sono state rilevate criticità che adesso le sintetizzo. Con il diploma ITS accademy, con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del quadro europeo delle qualifiche (EQF), il diplomato non può riscattare gli anni di studio ai fini pensionistici, come avviene per la laurea; può utilizzare al massimo solo 40 crediti formativi (CFU) del diploma biennale ITS (e non tutti i diplomi assegnano crediti) per proseguire un eventuale corso di studi, nella stessa area, in ambito universitario, mentre ogni anno universitario riconosce 60 CFU; non può utilizzare il valore legale del diploma per l'eventuale partecipazione a concorsi pubblici, che sono riservati o ai laureati o ai diplomati. Inoltre, i diplomi ITS non danno il titolo che dà una laurea triennale; ad esempio, il dottorato o qualcosa di similare. Capiamo bene che la *ratio* degli ITS è quella di formare personale da inserire subito in azienda, ma è lecito per un giovane cambiare idea o programma di vita dopo il percorso di studi, o magari anche, dopo avere lavorato, qualche anno dopo, quella formazione per passare ad altro lavoro. quindi, Ministro, se, nell'ambito del vasto lavoro che lei sta svolgendo a tal proposito, vi sia anche il superamento delle criticità appena indicate, anche d'intesa con gli altri Dicasteri competenti.

punto qualificante del PNRR per la componente istruzione, è scaturita dalla necessità di rendere la formazione terziaria professionalizzante più attrattiva per i giovani e di arricchire l'offerta formativa, anche in risposta alle esigenze del tessuto produttivo dei territori e delle nuove prospettive del mondo del lavoro e dell'economia. Ciò premesso, per l'attuazione della riforma il PNRR ha previsto un investimento di 1,5 miliardi. Per il riparto di queste risorse, il Governo ha avviato da subito un confronto con le Regioni, recuperando le distanze che si erano registrate in precedenza. Sono stati così subito ripartiti i primi 500 milioni per potenziare i laboratori già esistenti e realizzarne di nuovi, al fine di aumentare il numero di percorsi e incrementare le iscrizioni, con riserva del 40 per cento, negli ITS academy presenti nelle Regioni del Mezzogiorno. Inoltre, il 26 maggio scorso è stato approvato anche l'ulteriore decreto di riparto di 700 milioni di euro per incrementare l'offerta didattica e favorire una maggiore partecipazione delle aziende ai processi formativi. Quanto alle questioni specifiche poste dall'interrogazione, faccio presente che la legge di riforma n. 99 del 2022 estende già agli ITS academy la normativa in materia di riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici. In merito al collegamento più organico e strutturato tra il percorso della formazione terziaria non universitaria e il sistema terziario accademico, ricordo che la medesima legge prevede, a tale fine, l'adozione di un decreto interministeriale Mim-Mur. Sarà pertanto in quella sede che il Ministero punterà a valorizzare ed agevolare i passaggi tra ITS academy e università. Inoltre, relativamente al riconoscimento del valore legale del diploma per la partecipazione ai concorsi pubblici, la legge vigente prevede che i diplomi di quinto e sesto livello EQF costituiscano un titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Infine, con successivo decreto Mim-Mur sarà stabilita la tabella di corrispondenza dei titoli e dei crediti riconoscibili. Concludo rassicurando che questo Governo crede fortemente nell'attuazione della riforma degli ITS academy e che dunque agirà, anche attraverso i numerosi provvedimenti attuativi ancora previsti, affinché sia rafforzata l'attrattività di tali percorsi a beneficio dell'accrescimento delle competenze dei relativi studenti e al contempo a vantaggio della complessiva competitività del sistema produttivo del nostro Paese.

Sappiamo che il lavoro che sta svolgendo sul tema degli ITS academy è serio e che punta a massimizzare i risultati. Quindi, ci auguriamo che questo percorso di studi diventi un po' come quello già sperimentato negli altri Paesi, come la Germania, che ha dei percorsi universitari più teorici e altri più pratici. I giovani di oggi, come ho detto poc'anzi, hanno percorsi più duri dei nostri; dovranno cambiare lavoro più volte nella loro vita ed è opportuno che la formazione, i crediti formativi, le coperture previdenziali siano sempre adeguati e li accompagnino durante tutta la loro carriera. L'augurio è quello che vi siano tanti giovani che scelgano la formazione verso il mondo del lavoro, come quella degli ITS academy, ma che essi possano cambiare, se vorranno, conservando i propri diritti durante tutta la loro carriera.

Signor Presidente, signor Ministro, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, come lei ben sa, mette a disposizione del comparto scuola oltre 19 miliardi. Con l'obiettivo Scuola 4.0, gran parte di queste risorse sono destinate, non soltanto al rinnovo degli ambienti didattici innovativi, ma anche alla formazione digitale del personale, alla lotta alla dispersione scolastica ed anche all'aumento del tempo pieno pieno a scuola. Ora, alla data del 30 giugno 2023 è fissata la scadenza per l'entrata in funzione e l'utilizzo didattico dei laboratori per l'anno scolastico 2024-2025. Tuttavia, come lei ben sa, numerosi dirigenti e anche associazioni di categoria hanno sottolineato le notevoli difficoltà. Chiaramente, queste difficoltà sono date certamente dalla carenza di organico, certamente da una richiesta di proroga, in quanto impossibilitati a rispettare la scadenza stessa, e dalla mancanza di professionalità adeguate.

Inoltre, buona parte di queste risorse, come ben sa, è dedicata alla dispersione scolastica e abbiamo necessità che determinati decreti vengano emanati perché la dispersione scolastica, soprattutto in alcune parti parti del nostro Paese, è un *vulnus* davvero grave di cui dobbiamo occuparci. Abbiamo presentato questa interrogazione, quindi, per chiedere al Ministro se è a conoscenza di questa grave situazione e anche quali misure e iniziative intenda intraprendere per riuscire a far sì che queste risorse possano essere messe a terra per il mondo prezioso della scuola.

un'importante opportunità, come è stato ben detto, per la scuola italiana. In questi mesi, abbiamo lavorato molto per supportare le scuole, in molti casi risolvendo questioni frutto di errori di impostazione dello stesso Piano. Su tutti, cito i molteplici interventi in tema di semplificazione sia a beneficio delle scuole che degli enti locali. Inoltre, proprio per andare incontro alle esigenze e alle richieste delle istituzioni scolastiche, abbiamo individuato per loro percorsi di accompagnamento amministrativo per facilitare le procedure di affidamento. Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo incrementato la quota di acconto dal 10 per cento previsto dalle prime disposizioni del PNRR fino al 50 per cento proprio in considerazione della necessità, più volte rappresentata dalle scuole, di avere una maggiore disponibilità finanziaria iniziale. Posso comunicare anzi che proprio in questi giorni abbiamo iniziato a erogare le risorse relative al Piano scuola 4.0 e quelle relative alle azioni per il contrasto alla dispersione scolastica. Ciò dimostra che abbiamo ascoltato le esigenze delle scuole nei limiti delle regole e delle procedure stringenti del PNRR e abbiamo ogni volta trovato le soluzioni più efficaci. Da ultimo, voglio anticipare in questa sede che abbiamo appena accordato una proroga dei termini per l'affidamento dei servizi e delle forniture al 31 luglio 2023. Tale proroga contempera le esigenze delle scuole di avere un ulteriore margine temporale senza pregiudicare in ogni caso le relative *milestone* del PNRR. Desidero infine ricordare che in pochi mesi abbiamo ripartito nei tempi previsti importanti risorse a favore delle scuole sia per le STEM, con lo stanziamento di 600 milioni di euro, sia per la formazione del personale scolastico con 450 milioni di euro, nonché per il potenziamento dei percorsi Erasmus, raddoppiando le risorse annualmente disponibili; infine, altri 150 milioni sono stati stanziati per le competenze linguistiche.

Sono veramente contenta di avere contribuito con i Governi precedenti a far sì che adesso il suo Ministero abbia quasi 20 miliardi da poter investire nella scuola. Mi auguro che lei ne faccia buon uso.

significherebbe ulteriore dispersione scolastica e un regionalismo delle disuguaglianze. Glielo dico da docente che ha vent'anni di esperienza nella scuola italiana: se lavorerà bene per la scuola, noi saremo al suo fianco, ma basta proclami e cominciamo con le azioni concrete.

l'opposizione è stata espressa da UPI e ANCI e dalle Regioni che hanno sollevato preoccupazioni in merito agli effetti devastanti che avrebbe tale riforma che, a loro dire, comporterebbe l'accorpamento di molteplici istituzioni scolastiche con meno di 900 alunni; il dissenso si è tradotto nel mancato accordo in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni per la contrarietà di quattro Regioni, che tra l'altro hanno impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale, a cui si sono aggiunte anche Abruzzo e Sardegna, che hanno considerato la proposta irrispettosa verso le specificità dei territori e lesiva del diritto a un'istruzione di qualità; tra le criticità segnalate vi sarebbero anche la riduzione degli organici e la conseguente soppressione di scuole che penalizzerebbe soprattutto le regioni del Mezzogiorno e delle aree interne del Paese, con il rischio di aumentare le sperequazioni territoriali nell'erogazione del servizio pubblico essenziale garantito dalla Costituzione, ovvero la scuola; risulta agli interroganti che la norma non prevede chiusure di plessi scolastici né interviene sui criteri di formazione delle classi che continua ad essere regolata dal decreto del bensì conferisce maggiori margini di autonomia alle Regioni che possono procedere ad un'articolazione degli istituti scolastici a prescindere dal parametro rigido del numero di alunni minimo per singola istituzione scolastica,

e molto delicato. Innanzitutto desidero precisare che la grande maggioranza delle Regioni ha votato a favore della nostra proposta dimensionamento; aggiungo peraltro che la regione Abruzzo ha accolto favorevolmente i chiarimenti che noi abbiamo dato, quindi credo che da questo punto di vista il problema si sia risolto. In realtà noi stiamo attuando una

in Italia ci sono 40.000 plessi scolastici, cioè 40.000 edifici in cui ci sono insegnanti, studenti, banchi, arredi, personale; nessuno di questi 40.000 plessi scolastici verrà chiuso. Qui non si tratta di chiudere scuole, ma soltanto di razionalizzare

preside. Questo perché in Italia ci sono ben 860 reggenze, il che significa che lo stesso dirigente scolastico è costretto a fare due bilanci, due pubblicità di atti, due contrattazioni, eccetera. Noi andiamo ad eliminare le reggenze, a concentrare e a razionalizzare, facendo sì dunque che l'offerta sul territorio sia la più coerente possibile. Le risorse risparmiate saranno tutte reinvestite nella scuola, e questo è un primo punto. Non solo: proprio aver dato alle Regioni, al di là di qualsiasi numero prefissato, la possibilità di strutturare l'offerta sul territorio consentirà di tenere in considerazione le aree di montagna e le aree disagiate, e quindi di modellare la strutturazione delle istituzioni scolastiche a seconda delle esigenze dei singoli territori. la ringrazio. Ovviamente mi ritengo soddisfatta della sua risposta, che mi auguro possa definitivamente eliminare tutti i dubbi che sono stati sollevati in maniera pretestuosa circa il dimensionamento scolastico. Infatti tale dimensionamento, come lei ha sottolineato, produrrà una riduzione graduale nei prossimi dieci anni che interverrà solo sulle dirigenze scolastiche non sul numero dei plessi, che rimarrà invariato. Quindi non ci sarà la paventata chiusura di 700 scuole, bensì una riorganizzazione della dirigenza con l'eliminazione progressiva delle reggenze, che ovviamente comportano non solo problemi all'apparato amministrativo, ma anche a livello didattico, come anche tanti presidi hanno lamentato in questi anni. Questo per non parlare anche dello stress personale a cui viene sottoposto un dirigente scolastico. In tal modo ci sarà una una migliore programmazione pluriennale della rete scolastica e un miglioramento dell'efficienza amministrativa. Signor Ministro, la ringrazio ancora non solo per la risposta e per aver eliminato tutti i dubbi, ma anche per l'ottimo lavoro che lei sta portando avanti in un comparto così delicato e importante come la

Presidente, che mondo è quello in cui, se nasci donna, devi temere di morire ammazzata? È il mondo orribile in cui ha trovato la morte, con il suo bambino, Giulia Tramontano. Soprattutto, che mondo è quello in cui, se scompare una donna, nessuno pensa, almeno al primo impatto, che si sia potuta allontanare volontariamente o che abbia avuto un malore, ma si pensa immediatamente che qualcuno abbia potuto ammazzarla? È un mondo che ha normalizzato l'orrore; un mondo che conta il numero delle vittime come se si trattasse di un fatto ineluttabile di fronte al quale non possiamo fare nulla. Invece, signor Presidente, non è così. Noi possiamo e dobbiamo fare di più, partendo però da un presupposto irrinunciabile: abbiamo il dovere di riconoscere che questo fenomeno ha un carattere strutturale e affonda le sue radici in una cultura patriarcale che fa del corpo delle donne l'oggetto del possesso e del dominio altrui. È una cultura che non più tardi di un'ora fa, a proposito dell'uccisione di Pierpaola Romano, la poliziotta in servizio a Montecitorio, parlava di movente passionale. Signor Presidente, l'unico sentimento, quando viene ammazzata una donna, è quello di chi veramente l'amava e a queste persone in questo momento va il mio e il nostro pensiero.